L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Non so cosa gli abbia detto la testa a quest'uomo, ma sicuramente non lo ha voluto Fini, il suo capo, che ha dimostrato molta più intelligenza alla Camera di di Gasparri, che solo per notizia o per *gossip* (perché qui si va avanti a *gossip*) vuol far entrare - e lo ripeto - un criminale in quest'Aula. È una vergogna per l'Italia. È una vergogna che non faremo passare inosservata!

Pedica, la richiamo per la seconda volta. Lei ha parlato e non può impedirlo agli altri. E che questi due richiami siano messi a verbale, perché una cosa è manifestare le proprie opinioni,

Desidero manifestare il senso della mia indignazione per questa decisione dei Capigruppo. Penso che il Parlamento sia il luogo sacro della democrazia rappresentativa, in cui vengono anche simbolicamente rappresentati i grandi valori dei diritti umani, della democrazia, del rispetto di quei concetti che sono qui scolpiti nella nostra Aula: «Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà e a certezza del progresso civile fu proclamata la Repubblica italiana».

perché le Assemblee rappresentative siano il luogo in cui si promuove il rispetto di tali diritti. Certamente sono favorevole al dialogo ritengo che l'affermazione dei diritti dei popoli abbia bisogno di un dialogo, un dialogo tra Governi, tra personalità, ma non è possibile che nel luogo cardine della democrazia si faccia parlare un Capo di Stato che nel proprio Paese non garantisce quei diritti che la nostra Costituzione assicura. Quale lezione potrà darci il Capo di Stato della Libia? Quali indicazioni potremo ascoltare in silenzio, senza parlare anche a nome

Naturalmente ci sono altre sedi in cui è possibile mantenere aperti questi canali di dialogo, ma vi prego di non metterci nell'imbarazzo non metterci nell'imbarazzo di dover assumere comportamenti che manifestino, anche in occasione della visita del leader libico, il nostro profondo dissenso. Presidente, colleghi, innanzitutto vorrei invitare il senatore Pedica, se non gli dispiace, a portare rispetto nel momento in cui parla dei colleghi, perché o siamo tutti signori

perché credo che lei in quest'Aula qualche sceneggiata meno degna di un senatore l'abbia fatta. *(Commenti del senatore Pedica).* A parte tutto ciò, indubbiamente in Libia ci sono problemi di diritti umani.

facoltà. LONGO *(PdL)*. Signor Presidente, ammiro molto la coerenza del senatore Pedica, il quale, dopo avere tacciato un ospite in visita ufficiale in Italia

Se il tempio della democrazia, come dice il senatore Giaretta, è forte - come è forte oggi in Italia, nonostante i tentativi dell'Italia dei Valori di dire

che certamente può essere inviso a molti, che ha molta strada da percorrere, ma che ha già percorso una piccola strada verso una forma di democrazia in un Paese, la Libia, che, come sa il senatore Pedica,

sempre! PRESIDENTE. Presidente Belisario, lei non può difendere i comportamenti scorretti dei senatori del suo Gruppo. Lei deve aiutare la Presidenza a tutelare il diritto di tutti ad intervenire in quest'Aula, senza intolleranze e senza interferenze.

sull'obbedienza che si deve alle regole. Credo di aver finito. In realtà, per gran parte non ho capito perché, per fortuna mia, strutturale e culturale, certe cose dell'Italia dei Valori non le capisco e spero di non capirle mai a fondo.

che avevano supportato la decisione della Conferenza dei Capigruppo, nonché i precedenti, ovverosia in quali altre occasioni l'Aula del Senato ha ospitato Capi di Stato e autorità di livello internazionale. Non ho ricevuto risposta. Secondo mie ricerche personali, sicuramente suscettibili di imprecisioni, i precedenti si riferiscono a re Juan Carlos di Spagna e a Kofi Annan, Segretario generale dell'ONU.

Nella passata legislatura il Senato ospitò un'autorità morale di indubbio rilievo, come il Dalai Lama, certamente non nell'Aula del Senato, ma in altro luogo. altro luogo. Guardiamo con preoccupazione alla decisione della Conferenza dei Capigruppo e della Presidenza, una decisione che indubbiamente mette molti senatori in difficoltà. Chiedo di considerare l'appropriatezza della scelta dell'Aula del Senato per ospitare un Capo di Stato controverso per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, come appunto il colonnello Gheddafi.*(Applausi

interventi di un dittatore da balconi molto vicini ad una piazza che ha visto altri interventi di altri dittatori purtroppo appartenenti alla nostra storia.

io non devo esprimere qui una valutazione personale rispetto a tale decisione o a come ad essa si è addivenuti. I precedenti sono quelli che lei, senatrice Carloni, richiamava: in Aula hanno parlato re Juan Carlos e il Segretario generale

riferirò al presidente Schifani delle perplessità e delle valutazioni che qui sono state espresse. Circa i diritti umani, spesso il

l'unanimità al di là degli schieramenti di appartenenza. Penso che su questo tema e su come farlo pesare nella politica internazionale dei vari Paesi, dell'Italia come dell'Unione europea, ci sia da compiere

signora Sottosegretario, colleghe e colleghi, migliorare la salute e la protezione della mamma e del suo bimbo è uno degli otto obiettivi della campagna delle Nazioni Unite per eliminare la povertà estrema entro il 2015. L'Organizzazione mondiale della sanità, tramite la *partnership* per la salute materno-infantile, ha organizzato una serie di iniziative volte a ricercare fondi per finanziare azioni capaci di migliorare la salute materna nel mondo, tutto questo lavorando, ovviamente, con i Governi sia dei Paesi in via sviluppo, che dei Paesi più avanzati, e ieri abbiamo in quest'Aula analizzato molto bene che cosa significa intervenire direttamente e lo scopo utile per intervenire rispetto ai Paesi in via di sviluppo. Per questo il 23 gennaio - lo ricordavamo anche ieri - l'Organizzazione mondiale della sanità ha organizzato con l'associazione Osservatorio nazionale sulla salute della donna una riunione a Ginevra per discutere insieme gli obiettivi e le prospettive della salute materno-infantile anche in Italia, così come gli aspetti della politica estera, in merito a questo tema (di cui abbiamo parlato appunto ieri) e voglio ricordare anche oggi che la delegazione delle parlamentari parlamentari era formata dalle senatrici Boldi, Bianchi, Bianconi, Baio, Bugnano e Rizzotti e dalle onorevoli De Camillis e Paola Binetti. Tra l'altro, in quell'occasione l'Organizzazione mondiale della sanità ha insignito queste parlamentari del ruolo di consigliere temporaneo e questo, da una parte, è un grande onore, ma, dall'altra, anche una grande responsabilità. Attualmente la salute materno-infantile è ben presente nelle agende politiche delle Nazioni, ma c'è ancora molto da fare e la mozione di oggi indica anche quali sono le preoccupazioni e i punti di debolezza in Italia. Il tasso di mortalità materna è considerato come principale strumento per valutare lo stato di assistenza socio-sanitaria ed anche un indice importante per valutare il grado di sviluppo raggiunto da un Paese. Infatti, i 10 milioni di morti ogni anno legati al parto e alla prima infanzia nel mondo, che si potrebbero tutti prevenire, non sono certamente un dato confortante. In Italia, grazie alla nostra rete di protezione formata da professionisti e strutture adeguate possiamo fortunatamente non vivere questi drammi, ma i recenti dati ufficiali sulle nascite con taglio cesareo (rapporto Osservasalute del 2008) indicano una percentuale nazionale pari al 38,3 per cento, con picchi in alcune Regioni fino al 60

Le recenti statistiche dell'Unione europea indicano una media dell'Europa, ma per Nazioni, pari al 23,7 per cento: quindi, registriamo circa 15 punti in più rispetto alla media europea. Quelli degli Stati Uniti sono leggermente più alti perché si attestano intorno al 27,5 per cento. Su questi dati una riflessione va svolta su diversi campi. Intanto, esistono diversi fattori per spiegare questo fenomeno. Sono fattori clinici, il taglio cesareo andrebbe praticato solo in determinate circostanze. Anche per questo motivo, vi sono indicazioni molto precise e linee guida che andrebbero sicuramente tenute più presenti. Esistono poi fattori sociali. Uno dei fattori che potrebbe spiegare l'elevato tasso di parti cesarei è la richiesta da parte delle donne di utilizzare maggiormente questa modalità, sia per motivi di lavoro che di età. In alcuni casi questa domanda proviene dalle donne con età superiore ai 35 anni, che potrebbero quindi presentare anche gravidanze più rischiose.

visto che il parto dovrebbe essere un evento assolutamente fisiologico, nella normalità e soprattutto in situazioni non di patologia né per la madre né per il figlio, poi anche fattori sanitari. Il tasso di parti cesarei in Italia mostra una grande variabilità interregionale:

In tal senso - e devo dirlo per una attestazione di realtà, perché su queste tematiche non esiste centrodestra o centrosinistra - i Governi che si sono susseguiti hanno sicuramente messo in campo azioni molto importanti,

Questo, normalmente, è sempre il grande spauracchio delle Regioni e delle ASL. Il Comitato nazionale di bioetica ha stabilito nel 2001 che tutte le partorienti hanno diritto alla conoscenza delle tecniche per contrastare il dolore e nel 2006 è stato approvato dell'anestesia epidurale del parto tra le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale offre a tutte le donne. Il piano d'azione continua con la programmazione dell'allattamento al seno per promuovere la salute della donna, con un piano di vaccinazione contro l'HPV

promuovere, di concerto con le Regioni e le Province autonome, un appropriato ricorso al parto con taglio cesareo, attraverso l'utilizzo di strumenti informativi adeguati a rilevare tutte le informazioni possibili legate alla fase prenatale, all'evento nascita e al monitoraggio ad un anno

di promuovere l'appropriatezza del percorso nascita e della pratica clinica, tramite un'adeguata offerta dei punti nascita rispondenti a requisiti minimi strutturali e organizzativi per la promozione di protocolli per l'assistenza neonatale.

perché i loro Governi possano promuovere sempre più una protezione, una valorizzazione ed una conoscenza dei percorsi della salute materno-infantile in Italia e nel mondo. *(Applausi

Bianconi come l'Organizzazione mondiale della sanità raccomandi che i diritti umani delle donne, soprattutto quello alla salute, e i diritti sessuali ed alla riproduttività debbano essere protetti tramite politiche e programmi pubblici.

ed a questioni di carattere organizzativo delle nostre strutture sanitarie. Occorre che prendiamo atto una volta per tutte del disagio avvertito soprattutto tra le giovani donne, perché nel nostro Paese si continua a vivere il travaglio e il parto esattamente come nei secoli precedenti.

per cento ha potuto accedere all'anestesia locale o all'epidurale. Negli ultimi anni si è fatta strada anche nel nostro Paese l'idea dell'umanizzazione della cura e dell'ospedale senza dolore. È evidente che la lotta al dolore non può essere limitata solo ad alcune malattie particolarmente gravi, perché la filosofia che sottende all'eliminazione del dolore è legata al rispetto della persona e al valore del benessere come stato generale. La preoccupazione che vogliamo esprimere nasce dal fatto che, mentre non combattiamo con sufficiente decisione il dolore del travaglio e del parto, avanza a grandi passi una forma di medicalizzazione spinta della gravidanza, che rende la nascita un evento sempre più tecnologizzato. Cito alcuni dati a supporto di questa tesi: il numero medio delle ecografie effettuato durante la gravidanza è 5,5, quando il protocollo del Ministero della salute ne raccomanda al massimo tre; i parti effettuati mediante il taglio cesareo sono passati dall'11,2 per cento del 1980 al 38,36 per cento Vorrei ricordare che l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di rimanere tra il 10 ed il 15 per cento del numero dei parti totali, anche perché il conseguente aumento del numero dei parti cesarei significa anche un aumento da due a quattro volte del rischio di mortalità materna.

quello organizzativo, giacché il ricorso al parto cesareo appare più diffuso nelle strutture private; quello comportamentale, proprio per la diversità dei comportamenti del personale sanitario, che evidentemente non è in rapporto ai livelli di appropriatezza che dovrebbero essere ampiamente condivisi. Inoltre manca quello dell'informazione, necessaria per consentire alle donne di vivere in piena consapevolezza la gravidanza ed il parto. È molto limitata infatti la possibilità di frequentare i corsi di preparazione al parto e, anche in questo caso, vi sono forti differenze geografiche:

La preparazione al parto è uno dei fattori decisivi per affrontare in modo informato e corretto la maternità e anche per favorire la salute della madre e del bambino, ma serve anche per rafforzare il senso della genitorialità,

negli ultimi anni abbiamo assistito ad una costante riduzione della rete dei consultori e delle loro funzioni, in particolare in alcune Regioni; c'è anche un evidente parallelismo tra la minore presenza di questi servizi materni ed infantili nel Sud e nelle isole ed un maggiore tasso di mortalità neonatale ed infantile; in queste Regioni, poi, sono più numerosi i bambini che nascono sotto peso e si ricorre molto meno all'allattamento al seno. Sono tutti fattori che incidono negativamente sulla salute delle madri e dei bambini. Nella precedente legislatura, con il Governo Prodi, era stato presentato alla Camera un disegno di legge di iniziativa governativa, il n. 1923, che aveva per titolo «Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato» che tuttavia non ha potuto essere approvato a causa dell'interruzione della legislatura stessa. Inoltre, si era aperto un dibattito tra le componenti delle Commissioni parlamentari sulla inadeguatezza dei servizi di assistenza al parto.

comma 3, che «Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale nelle strutture individuate dalle regioni e all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse»; Nel giugno 2008 c'è però stato riferito dal ministro Sacconi che questi livelli essenziali di assistenza, non essendo finanziati, non sono applicabili sappiamo che su una modifica dei LEA si è aperto un tavolo con le Regioni. Una cosa è chiara: se i LEA non saranno finanziati, le donne continueranno a partorire con dolore e a ricorrere, anche quando sarebbe evitabile, al parto cesareo, con costi per il Servizio sanitario nazionale ben più elevati rispetto all'espletamento di parti naturali con l'utilizzo dell'epidurale.

per il sollievo dal dolore che in determinate realtà è completamente assente; a verificare i dati sulla morbilità e mortalità materna e neonatale e ad effettuare una rilevazione dei costi relativi a tale pratica e un censimento delle strutture abilitate; a promuovere campagne informative volte a rendere più consapevoli delle proprie scelte le donne che ricorrono al parto cesareo; a promuovere un'appropriata assistenza alla nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante; assicurare la tutela della salute materna, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità; a ridurre i fattori di rischio di malattia pre e postconcezionali del nascituro attraverso appropriati interventi preventivi; potenziare l'attività dei consultori familiari, ad assicurare la qualità dell'assistenza ostetrica e pediatrico-neonatologica nel periodo perinatale; contrastare le disparità territoriali e sociali in ordine all'accesso ai servizi per la tutela materno-infantile, anche per la popolazione immigrata vorrei chiedere di prevedere l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria e di mediazione culturale per le donne immigrate; promuovere l'offerta attiva di informazione e di consulenza alle donne prima della gravidanza, alle gestanti e alle puerpere, anche mediante corsi di accompagnamento alla nascita; favorire il controllo e la gestione del dolore nelle fasi del travaglio, nel quadro di una maggiore e migliore umanizzazione dell'evento nascita, anche attraverso il ricorso a tecniche avanzate di anestesia locale e di tipo epidurale. Signor Presidente, queste sono le questioni che chiediamo di porre al centro del nostro dibattito, ma anche di una politica precisa da parte di questo Governo che

*(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustro sinteticamente la mozione presentata dal mio Gruppo sul tema del parto cesareo. In Italia i dati statistici ufficiali più recenti, relativi alle nascite operate con taglio cesareo, ricostruiscono una situazione singolare nel panorama dei Paesi occidentali. Nel nostro Paese infatti i tagli cesarei hanno raggiunto percentuali superiore al 35 per cento del totale, con una percentuale vicina o superiore anche al 50 per cento in alcune Regioni, soprattutto nel Sud Italia, quali Campania, Basilicata, Sicilia, Molise, Puglia, Abruzzo e Calabria. Inoltre, in diverse cliniche operanti in grandi città italiane, come Roma, le percentuali relative ai parti con taglio cesareo raggiungono valori vicini all'80 per cento del totale; al contrario, analizzando i dati relativi alle Regioni settentrionali, si scorgono valori, seppur in aumento, di gran lunga inferiori al dato medio nazionale. Analizzando i dati relativi al Continente europeo si registra un fenomeno similare di forte crescita, ma si evidenzia una netta differenza con le percentuali riscontrate in Italia; in Europa, infatti, il dato medio ufficiale non raggiunge il 30 per cento l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte reso noto che solo il 10-15 per cento delle gravidanze dovrebbe sfociare in un parto cesareo, ovvero ciò dovrebbe accadere nei casi di donne con un posizionamento dell'utero anomalo, con *herpes* genitali, o con qualsivoglia altro impedimento che giustifichi la scelta dell'operazione chirurgica sulla parte uterina ed addominale; in circostanze di elevato rischio per le madri o per i nascituri la scienza medica non ha mai avanzato dubbi sull'utilità del parto cesareo, ma al contempo occorre ricordare che il parto vaginale è la modalità normale e più corretta per portare a termine una gravidanza; anche perché nella maggior parte dei casi le donne che partoriscono con il cesareo devono affrontare un ricovero più lungo, a volte più doloroso ed un rischio più alto di infezioni. inoltre, da studi recenti non ancora con evidenza scientifica, che i bambini nati con parto cesareo abbiano una maggiore probabilità di soffrire di asma, dovuta alla mancata esposizione ai batteri della mamma, cosa che accadrebbe, invece, nel parto naturale e che provoca lo sviluppo di difese immunitarie più forti. Infatti, analizzando i dati dei parti cesarei programmati prima della trentanovesima settimana, si notano alte percentuali di rischio di problemi respiratori per il neonato. Purtroppo, spesso la tendenza a preferire il parto con taglio cesareo non avviene per particolari indicazioni cliniche, ma per esigenze organizzative dei medici e delle stesse donne. Molti medici optano per il taglio cesareo in ragione del fatto che l'operazione e l'anestesia sono diventate più sicure che in passato, sebbene non vi sia prova che indichi che la gravidanza ed il parto vaginale siano più pericolosi che qualche decennio addietro, o anche perché applicano una sorta di medicina difensiva da eventuali denunce o più in generale da accuse relative a complicanze non classificabili come errori. In assenza di complicazioni di tipo medico, per la donna come per il nascituro, il parto vaginale è quello che garantisce una miglior ripresa dopo il parto stesso, permettendo successivi parti in tempi ristretti. Dal 2007 in poi molte strutture d'avanguardia in Italia hanno ridotto il numero dei parti cesarei grazie all'offerta sempre più ampia di anestesia epidurale. Poiché è compito dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Costituzione, garantire la salute della popolazione e, inoltre, l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda da sempre la protezione del diritto alla salute tramite politiche pubbliche di attenta programmazione, la mozione impegna il Governo a promuovere, di concerto con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, soprattutto nelle Regioni in cui i dati hanno evidenziato un aumento spropositato dei parti con taglio cesareo, campagne informative volte a rendere più consapevoli delle proprie scelte le donne che optano per il parto cesareo; ad eliminare eventuali tendenze dei medici a favorire il tipo di parto più remunerato in luogo di quello naturale, o comunque più indicato per il benessere della donna e del neonato; a promuovere iniziative legislative per limitare il fenomeno del condizionamento dei medici, dovuto ai rischi penali connessi allo svolgimento del proprio lavoro, nella scelta dei trattamenti da intraprendere; ad emanare linee guida contenenti indicazioni specifiche sull'opportunità di preferire il parto naturale, quando non pericoloso per la salute della madre o del bambino; promuovere l'inizio immediato dell'allattamento, favorendo un'educazione della madre nel periodo preparto; assicurare, per il benessere psicologico della donna partoriente, la presenza di una persona, familiare o non, di sua scelta durante il parto; infine, promuovere e garantire l'anestesia epidurale gratuita. Vi

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici, senatori, onorevole sottosegretario Roccella, le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di gravidanza e parto informano che non c'è alcuna giustificazione, in nessuna regione geografica del mondo, per avere più del 10-15 per cento di parti cesarei. In ogni luogo l'Organizzazione mondiale della sanità afferma che non c'è alcuna prova avvalorata scientificamente che dopo un primo cesareo sia necessario un ulteriore cesareo per la gravidanza successiva. Sono nozioni che appartengono ad un'altra quella in cui io studiavo medicina all'università, gli anni Settanta, in cui la regola che si sosteneva era «una volta fatto un cesareo, sempre cesareo». Oggi i dati della letteratura scientifica dicono che la probabilità di rottura dell'utero in donne con una singola incisione trasversa del segmento inferiore dell'utero

dagli anni Ottanta agli anni Novanta. La realtà nel nostro Paese va purtroppo nella direzione opposta. In Italia si registra il più alto numero di cesarei in Europa e vantiamo il secondo posto nel pianeta, dopo il Brasile. tuttavia sottolineata una differenza marcata tra le varie Regioni con situazioni davvero difficili da giustificare: in Campania si ricorre al cesareo nel 60 per cento dei parti, in Basilicata nel 54,4 per cento, in Sicilia nel 52,4 per cento. Non possono essere solo le motivazioni mediche a giustificare questi numeri, ma ormai la prassi la prassi è talmente consolidata e radicata anche sotto il profilo culturale che molte donne preferiscono il taglio cesareo; addirittura lo chiedono perché sono convinte erroneamente che si tratti di un parto più sicuro. Sono credenze che non hanno alcun fondamento, dato che il rischio di mortalità materna per cesareo è di tre-quattro volte superiore rispetto al parto vaginale: chi mi ha preceduto ha sottolineato molto bene che si tratta di Inoltre, non è nemmeno paragonabile il tempo di recupero dopo il parto per una donna che ha subito un taglio chirurgico, che spesso non riesce ad alzarsi dal letto prima di ventiquattr'ore e a tenere in braccio il proprio bambino. La degenza media è infatti superiore e la donna deve rimanere in ospedale tre o quattro giorni invece di tornare a casa

Il fenomeno è noto, ma fino a questo momento non vi è stata alcuna politica di intervento efficace per tentare di ridurre il numero dei cesarei, perlomeno nelle Regioni del Meridione. Si parla di fattore geografico e di fattore organizzativo. Questo significa che si ricorre maggiormente al cesareo nelle Regioni del Sud, dove ci si rivolge frequentemente alle strutture private accreditate.

basata solo su valutazioni cliniche è confermato dal fatto che negli ultimi anni in Italia i parti naturali sono aumentati significativamente nelle Regioni che hanno introdotto dei meccanismi di incentivazione

cesareo non è quasi mai la prima opzione per una donna, ma una soluzione accettata nel momento in cui il medico la prospetta come migliore e più sicura. È invece importante che la donna abbia la consapevolezza che il parto naturale è sempre l'opzione migliore, così come lo è l'allattamento al seno e la presenza del bambino nella stanza con la mamma dal momento del parto e per tutta la durata della permanenza in ospedale o nella clinica. Spesso nella richiesta da parte delle donne di sottoporsi al taglio cesareo vi è anche una seconda componente psicologica molto comprensibile, che riguarda la paura del dolore nella fase del travaglio. Questo aspetto potrebbe essere facilmente affrontato con risposte concrete, se solo si fornissero su tutto il territorio nazionale le risorse necessarie ad un parto indolore. Le tecniche esistono e sono ormai largamente diffuse e consolidate. Vengono usate, per esempio, in Paesi come la Gran Bretagna e la Francia nel 70 per cento dei parti e negli Stati Uniti la percentuale in Italia purtroppo siamo fermi, con i dati del 2001, al 3,7 per cento. In alcune Regioni per poter eseguire il parto con l'epidurale ci si deve allontanare di centinaia di chilometri e in altre il servizio viene assicurato solo a pagamento. Per concludere, vorrei sottolineare che con la mozione che presentiamo oggi, illustrata dalla senatrice Bassoli, chiediamo che il Governo si impegni a fare un serio e costante monitoraggio dei parti cesarei,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, a partire dalla fine degli anni Cinquanta abbiamo assistito indubbiamente ad un progressivo aumento dei parti cesarei e quindi ad una progressiva confluenza dell'evento nascita verso le strutture ospedaliere. La nascita per secoli, storicamente, è stata una presenza quotidiana nella vita sociale, un momento impegnativo, ma che era vissuto da intere famiglie in modo unitario e con una *affectio* particolare. Tutti erano protagonisti al momento della nascita di un bambino, non solo la mamma e il bambino ma intere famiglie. Il progressivo aumento dei parti cesarei

a dimenticare le sensibilità del neonato e della partoriente ed a far sì che la donna svolga poco più che un ruolo passivo nella nascita del proprio figlio. Le motivazioni sanitarie che forse vi erano qualche tempo fa e che erano sostanzialmente legate a precarie condizioni igienico-sanitarie

procreare naturalmente sono legate sostanzialmente all'età della donna, che molto spesso ha posticipato il momento in cui

nel momento della nascita del figlio, cioè al fatto che il figlio non rischi nulla nel momento in cui nasce.

di tipo diverso. Possiamo dire tutti che il parto è l'esperienza più alta della vita della donna e sicuramente anche del padre, quindi dell'uomo:

Per facilitare parti fisiologici e nello stesso tempo venire incontro alle esigenze di quelle donne che hanno una soglia di sofferenza più bassa o non si sentono di affrontare il dolore nel momento del parto, credo sia

Signor Presidente, mi deprime intervenire oggi su questa tematica: la depressione non sarà una categoria politica, ma esprime il senso di disagio di una donna italiana che nel 2009 deve affrontare il tema dell'essere donna in Italia.

abbiamo le leggi più violente che entrano nel nostro corpo, come la n. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita; stiamo negando perfino l'accesso all'aborto farmacologico, perché solo quello chirurgico può criminalizzarci meglio; e stendiamo un velo pietoso sull'aborto terapeutico. Siamo ancora qua, con alcune mozioni, ad affrontare temi come quello dell'abuso del ricorso al taglio cesareo, che va ovviamente in coppia ed è una conseguenza della negazione del parto senza dolore. Troppo facile il richiamo al rispetto letterale del precetto biblico «partorirai con dolore»: troppo facile e semplice. Non basta, e c'è di più.

e i LEA (poi scomparsi). E allora torno, per concludere, alla mia depressione politica e personale di donna italiana che, solo grazie

urlavano e molte ancora oggi continuano ad urlare e a vedere per la prima volta il loro figlio in un bagno di lacrime che spesso le fa desistere dall'avere un secondo figlio.

l'Italia effettivamente detiene oggi quasi il primato di parti cesarei nel mondo occidentale, con il 38,3

soprattutto nelle cliniche private, dove 6 bambini su 10 nascono con il parto cesareo. Ciò che fa veramente specie è che, almeno nel 50 per cento di di quei casi (è testimonianza delle partorienti), non viene nemmeno spiegato chiaramente il motivo per cui si ricorre al parto cesareo. Questo naturalmente quando, come è stato già illustrato da altri colleghi, non è la donna stessa che chiede il cesareo per svariati motivi: la paura di un parto naturale, il fatto di voler programmare la nascita o di ritenere che il bambino corra meno rischi. In realtà, credo rischi. In realtà, credo sia abbastanza ingiusto allontanare le donne dal parto naturale anche perché nel tempo vi è il rischio assoluto di aumentare ulteriormente nelle donne la paura del parto.

che ultimamente sia passato il concetto che la gravidanza non sia un fatto naturale ma uno stato di malattia, cosa che non è nel modo

minacciose che non credo corrisponda al vero. Le vere gravidanze a rischio, in realtà, sono molto ridotte percentualmente rispetto alla quantità totale delle gravidanze. Chiaramente dalla gravidanza a rischio si passa alla necessità del parto cesareo. Questo è un non senso perché sappiamo invece che il parto cesareo ha

è a tutti gli effetti un intervento chirurgico, con tutto quello che qualunque intervento chirurgico porta con sé. Quindi, potremmo

alcune Regioni meridionali, come la Campania e la Calabria, il ricorso al parto cesareo è maggiore, questa va ricercata anche nella non efficienza di

darebbe anche una spiegazione del motivo per cui, soprattutto nelle strutture private, si preferisce il ricorso al parto cesareo. Fino a quando ci sarà un rimborso economico maggiore

Credo rischi di più quando, per qualche motivo, non ha fatto, come doveva, tutte le valutazioni necessarie prima di arrivare al parto. Ad esempio, nelle nostre cliniche universitarie di ostetricia e ginecologia non si insegna più a fare la valutazione del rapporto feto-pelvico, che non necessita di alcuno strumento particolare, ma semplicemente di un esame di tipo semeiologico. Non si insegnano più tantissime cose che prima si insegnavano e, dirò di più, più, si insegnavano addirittura ai medici generici, neanche agli ostetrici e ai ginecologi specialisti: ricordiamoci che in Italia per tantissimo tempo c'erano i medici condotti che erano in grado, benissimo, di far partorire le donne. Ora è giusto che non si segua più

anche in un'Aula parlamentare. Infatti, anche dall'approvazione di queste mozioni, nonché dalla collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con la *partnership* dell'OMS,

Signor Presidente, sempre più spesso Senato e Camera discutono e approvano mozioni che fanno riferimento alla salute delle donne spingendo all'assunzione di un punto di vista di genere nella pratica medica e nell'organizzazione della sanità pubblica e sempre più spesso tali mozioni incontrano e sollecitano un interesse che supera ogni logica di parte e che insiste sulla necessità di innovazione, sia scientifica sia gestionale, perseguendo il benessere delle persone, in questo caso delle donne e dei nuovi nati. È il caso delle mozioni che oggi stiamo discutendo, che parlano tutte lo stesso linguaggio. Con riferimento particolare alla mozione che vede come prima firmataria la senatrice Bianconi, vorrei esprimere il mio apprezzamento e la speranza che il Governo, conseguentemente, assuma le indicazioni proposte, a cominciare appunto dalla diffusione del sistema analgesico peridurale di cui tanto si è discusso. La mia Regione, la Campania, ha in Italia il primato negativo del ricorso al parto cesareo. Tutti i dati in nostro possesso fanno registrare un eccesso di medicalizzazione dell'evento nascita. La percentuale di nati con taglio cesareo, pari al 63 per cento, non è certo spiegabile con specifiche caratteristiche delle partorienti o dei neonati napoletani. Inoltre, il ricorso al taglio cesareo è meno frequente nelle strutture pubbliche, come è stato qui detto, rispetto a quelle private. Nel caso campano, però, e nel caso delle private il dato è pari al 72,6 per cento e qui, paradossalmente, si concentra la maggioranza dei parti a più basso rischio. Le caratteristiche di questa vera e propria epidemia, che ha visto una crescita esponenziale del fenomeno (passato dal 20 per cento del 1990 al 61,5 per cento sono tali da avere sollecitato allarme e reazione a vari livelli, a cominciare dalle *élites* femminili più consapevoli e dagli operatori sanitari più responsabili. In questi anni è cresciuta una forte volontà di contrasto, che ha trovato il suo centro propulsore nell'attività della dirigenza femminile della Regione Campania e nelle iniziative della giunta.

certamente ancora non significativa al fine di aggredire e abbattere una *malpractice* di proporzioni così importanti. Tuttavia, mi interessa portare all'attenzione un fatto reale e cioè che, finalmente, l'azione di contrasto da parte del governo regionale è sistematica, coerente e determinata e che si è almeno interrotto un ciclo di crescita esponenziale. Quanto accade è che, almeno una volta all'anno, in occasione della pubblicazione del rapporto sulla natalità e nati-mortalità in Campania per iniziativa della Regione, il tema è portato all'attenzione della pubblica opinione sottoponendo l'azione degli amministratori pubblici a verifiche stringenti nel raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida regionali. Infatti, dal dicembre 2007, la Giunta si è dotata di un atto di indirizzo per la promozione del parto fisiologico che migliorava e rafforzava precedenti linee guida per la riduzione dell'incidenza del parto cesareo, anche alla luce di un pronunciamento di sospensiva del TAR Campania sulle metodologie sanzionatorie di regressione tariffaria tariffaria adottate in precedenza dalla Regione per quelle prestazioni di ricovero per parto cesareo che più clamorosamente si scostavano dagli standard nazionali. Il nuovo atto assume, diversamente, un sistema di disincentivi più appropriato sulla base di indicatori e codici di rischio ampiamente validati. Se però è vero che misure di disincentivo economico sono importanti, tuttavia abbiamo ben chiaro che da sole esse non fanno una strategia vincente. Infatti, l'epidemia campana non è riconducibile esclusivamente al sistema dei DRG, ai rimborsi ed alla fame di cassa. È ovvio che questi interventi dall'alto non bastano a risolvere un problema che è anche culturale e che si lega alle carenze organizzative e strutturali strutturali note. Occorre quindi intervenire prioritariamente per dare alle donne un'informazione corretta. A questo proposito, un dato critico molto significativo è quello che vede solo una gestante su dieci partecipare ai corsi preparto. L'informazione alle donne, l'impegno di tutti gli operatori nei centri nascita (a cominciare dalle ostetriche oltre che dai ginecologi), la discussione, la valutazione e la diffusione di pratiche efficaci, l'apertura di case di maternità (cui si sta provvedendo), il ruolo dei consultori, il potenziamento del sistema informativo sulla natalità e una strategia integrata in tal senso costituiscono le chiavi di volta di una realtà certamente grave,

come è già stato detto, l'Italia è il Paese con il più alto numero di parti con taglio cesareo dell'Unione europea. I risultati delle indagini confermano un incremento dei numeri dei numeri relativi alla quota dei cesarei che, pure aumentando in modo generalizzato su tutto il territorio, raggiunge livelli particolarmente elevati nell'Italia meridionale e insulare. L'incidenza di parti cesarei, come è stato già detto, è particolarmente alta nelle strutture private rispetto a quelle pubbliche. Fondamentali per ridurre il ricorso improprio al taglio cesareo sono una corretta valutazione del rischio e la promozione di specifici percorsi assistenziali differenziati per il profilo di rischio. La tutela della maternità va affrontata attraverso l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscano alle donne di essere salvaguardate sia nel momento in cui affrontano la gravidanza, sia quando affrontano i problemi connessi al parto. Occorre contrastare le disequità territoriali e sociali di accesso ai servizi per la tutela materno-infantile anche per la popolazione immigrata attraverso l'adozione di modelli basati sull'offerta attiva, migliorando la fruibilità dei servizi da parte della popolazione più svantaggiata e prevedendo l'attuazione di programmi di assistenza socio-sanitaria di mediazione culturale per le donne immigrate e una specifica intesa con le Regioni. La corretta valutazione dei rischi in cui incorre la donna nel corso della gravidanza ed in occasione del parto rappresenta la base per una valida impostazione di un piano di assistenza appropriato e per la precoce individuazione delle potenziali complicanze. Pertanto, occorre provvedere alla classificazione del rischio al momento del ricovero a cui devono conseguire specifici percorsi assistenziali differenziati per profilo di rischio. La valutazione del profilo deve essere effettuata sulla base di criteri (fattori biologici, sociali, psicologici) condivisi dall'*équipe* assistenziale (ostetrico, ginecologo, neonatologo, anestesista ed eventuali altri specialisti coinvolti nell'assistenza della gestante) e accuratamente riportati nella documentazione clinica. Deve, inoltre, essere caratterizzata da un processo di rivalutazione continuo e dinamico che non può in ogni caso sostituire un'adeguata e continuativa sorveglianza della donna e del feto nel

clinici, valori così elevati non sembrano giustificati da una maggiore frequenza delle condizioni cliniche (ritardo di crescita intrauterina, patologie della placenta, sproporzione feto-pelvica, gravidanze multiple ed altro) che, correttamente, possono rappresentare un'indicazione ad assistere il parto con taglio cesareo. Importante è poi il contesto sociale, culturale e sanitario nel quale la donna vive la sua esperienza riproduttiva. L'aumento di età delle donne alla nascita dei figli incide sul loro comportamento nel corso della gravidanza. Tra le donne che decidono di avere un figlio in una fase avanzata della vita si registra un più elevato livello di informazione e una maggiore capacità di autodeterminazione sulle scelte da compiere durante la gravidanza e al momento del parto. Non di meno, gli stessi fattori sono alla base di un'eccessiva medicalizzazione e di un sovrautilizzo delle prestazioni diagnostiche, che rischiano di trasformare gravidanza e parto da eventi naturali in eventi patologici.

Le Regioni meridionali e insulari presentano dati peggiori di quelle centrali e settentrionali per quanto concerne il ricorso al parto cesareo e all'anestesia generale, il tasso di mortalità neonatale e infantile, il basso peso alla nascita, il ricorso all'allattamento al seno. Nell'ambito di tale concentrazione geografica, si evidenzia tuttavia un fattore organizzativo costituito dalla maggiore diffusione del taglio cesareo nelle strutture private accreditate con particolare criticità in quelle della Campania. Campania. Altrettanto importanti sono poi i fattori sanitari costituiti dalla variabilità del comportamento dei singoli medici anche operanti in simili condizioni organizzative o, a volte, nella stessa struttura sanitaria; dalla relazione medico-paziente-*équipe* sanitaria; dalla completa informazione e preparazione che il personale sanitario fornisce alle pazienti; dalla eccessiva medicalizzazione del percorso nascita. Non tutti gli ospedali possono fornire un livello di sicurezza e non tutto il personale ostetrico è disponibile ad affrontare un aumento del rischio. Dato che la maggior parte degli ospedali non tutelano il medico in caso di complicazioni, i medici preferiscono il cesareo per evitare problemi legali nel caso si verificasse qualche complicazione e inconveniente durante il parto. Potrebbe esistere una correlazione tra i tassi elevati e l'inadeguatezza delle strutture sanitarie nelle Regioni. Il primo cesareo rende più a rischio la donna che incorre nella seconda gravidanza, secondo un pensiero ormai largamente abbandonato, costringendola per i parti successivi ad altrettanti cesarei. C'è comunque un incremento della richiesta materna di taglio cesareo, nonché un incremento di gravidanze da tecniche di procreazione medicalmente assistita che, di conseguenza, porta un incremento di gravidanze multiple. La gravidanza multipla implica, comunque, un'indicazione al taglio cesareo. Non ultimo, le assicurazioni private rimborsano il parto con taglio cesareo ma non le spese di parto naturale. La realtà è che il parto, a differenza della gravidanza, fa un po' più paura a tutte le donne, sia a quelle che partoriscono per la prima volta che a quelle che sono già mamme. Mentre la gravidanza rientra tra quei fenomeni vissuti in modo soggettivo da ciascuna donna, il parto per alcune può diventare un pensiero fisso per tutto il tempo della gravidanza e in questo caso poter utilizzare l'anestesia peridurale renderebbe sicuramente le donne più serene. Un clima di maggiore serenità indurrebbe qualsiasi futura mamma ad evitare condizionamenti da racconti altrui o retoriche da copertina. Un parto naturale, a differenza di un cesareo, consentirebbe di proseguire il normale corso della natura non solo nella gestazione ma soprattutto fino alla sua conclusione e, quindi, alla nascita, ove possibile naturalmente, quando non ci sono motivi e criteri che dettano veramente l'intervento chirurgico. Infatti, il parto cesareo è un evento traumatico come qualsiasi altro intervento chirurgico e, come tale, andrebbe evitato se non strettamente necessario. Il cesareo dovrebbe essere consigliato e adottato solo per motivi di necessità e urgenza o all'insorgere di complicazioni. Pertanto, credo che il Parlamento ed il Governo abbiano il dovere di intervenire presso le Regioni per cercare di arginare questa tendenza delle donne italiane al ricorso al parto cesareo, informandole anche su altre tecniche che inducono il parto naturale e presentando tutti gli aspetti determinanti nella scelta che ogni gestante è chiamata a fare al momento del parto, fornendo ogni elemento utile a valutare bene e soprattutto capire quando il cesareo è davvero necessario e quando invece è meglio addirittura evitarlo. Dopo una corretta informazione e una seria assistenza alle donne, le stesse donne, sentiti i consigli e i suggerimenti di quanti le assistono, potranno liberamente e più serenamente scegliere come partorire, fatti salvi, ovviamente, i casi di urgenza e di necessità o l'insorgenza di complicanze in cui tale libera scelta non può essere attuata. Perciò, proprio per consentire al Governo di adottare tutti i provvedimenti che possono garantire alle donne di essere salvaguardate, sia quando affrontano la gravidanza sia quando devono tutelare il loro diritto alla vita e ad una maternità serena e responsabile, ritengo assolutamente inderogabile convenire con i richiami contenuti nelle mozioni che stiamo esaminando. Tutte le donne andrebbero preservate da implicazioni o rischi che possono intervenire in prossimità del parto e ciò dovrebbe avvenire in maniera non difforme sul territorio nazionale, senza differenziazioni tra diverse aree del Paese. Dovremmo riuscire a divulgare le tecniche e le tradizioni migliori laddove ancora non ci sono, anche in tema di preparazione al parto. Allo stesso modo i medici dovrebbero avere tutti la stessa sensibilità, al Nord, al Sud, come al Centro e nelle Isole, ed essere in grado di praticare uniformemente in Italia, e non di meno eticamente ed efficacemente, le stesse pratiche diagnostiche e terapeutiche di documentata efficacia e di estrema attualità per la sanità pubblica, per la salute delle donne e quella dei neonati. Non è più tollerabile, infatti, che una donna, a parità di condizioni cliniche, possa ricevere cure differenti e partorire in maniera differente a seconda del luogo presso il quale viene assistita. Occorre contrastare fortemente le disequità territoriali e sociali di accesso ai servizi per la tutela materno-infantile per tutte le donne italiane ma anche per le donne immigrate, per garantire a tutte l'adozione dei medesimi modelli assistenziali. In conclusione, per ridurre il ricorso improprio al cesareo, sarebbe necessario costituire un gruppo multidisciplinare composto da ostetrici, ginecologi e ricercatori in sanità pubblica e, secondo la guida del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, predisporre linee guida cliniche italiane

da distribuire presso consultori, ambulatori pubblici e privati, corsi preparto e quant'altro. Sono infatti convinta che un buon livello di informazione, oggi ancora limitato, non potrà non indurre ciascuna donna in stato di maternità a fare le scelte migliori per sé e per il suo bambino.

temi, come quello della maternità, che raramente vengono affrontati nelle Aule parlamentari e che invece dovrebbero essere senz'altro esaminati. Infatti, se vogliamo dare concretezza all'idea del valore sociale della maternità, non possiamo tenerli lontani dal cuore della politica. La tutela della maternità e la promozione dell'appropriatezza del percorso nascita costituiscono per il nostro Ministero un impegno di valenza strategica, che si è già concretizzato in numerose iniziative. Tra le cause della crescita esponenziale del ricorso al parto cesareo negli ultimi 15 anni vanno certamente comprese l'eccessiva medicalizzazione della gravidanza e la sovrautilizzazione delle prestazioni diagnostiche nella gravidanza fisiologica come conseguenza indiretta dell'impoverimento dei saperi femminili e della competenza materna. Penso, ad esempio, alla difficoltà con cui si è tornati all'allattamento al seno, oggi raccomandato da tutti gli organismi internazionali, dopo che negli anni Cinquanta era stato fortemente promosso dalla classe medica l'allattamento artificiale; penso anche ad una visione dell'emancipazione femminile non come valorizzazione della differenza, ma come un appiattimento sul modello maschile

L'aumento del ricorso al taglio cesareo si registra soprattutto tra le donne di età avanzata e tra quelle che partoriscono nelle strutture sanitarie private. In merito all'eccessivo ricorso a prestazioni diagnostiche in gravidanza, presso questo Ministero è attualmente operante un tavolo tecnico, istituito al fine di verificare l'applicazione del decreto del Ministro della sanità 10 settembre 1998, di aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995. Nell'ambito dei lavori sono state formulate anche alcune proposte di modifica degli allegati A e B del medesimo settembre 1998 (riguardanti gli accertamenti in gravidanza esenti da ticket), che seguono le più recenti evidenze scientifiche, in sintonia con le linee guida sulla gravidanza fisiologica che stanno per essere predisposte da un *panel* di lavoro presso l'Istituto superiore di sanità (dovrebbero uscire ad ottobre). L'approccio ad un problema di natura così complessa prevede quindi interventi multipli, con una sinergia tra diversi attori istituzionali e professionali, allo scopo di promuovere interventi di sanità pubblica finalizzati al contenimento del fenomeno e al recupero dell'appropriatezza della pratica clinica. Al riguardo è in corso di predisposizione presso questo Ministero, in attuazione dell'articolo 79 del decreto-legge n. 112 del 25 con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, un decreto ministeriale finalizzato all'individualizzazione da parte delle Regioni delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza. È fondamentale ricordare l'accordo del 25 marzo 2009 sancito da Governo e Regioni che definisce gli obiettivi del Piano sanitario nazionale 2009, con cui si promuove l'appropriatezza del percorso nascita favorendo il parto naturale, con la garanzia per ogni parto dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ostetrica e pediatrica-neonatologica e della massima corrispondenza tra necessità assistenziali della singola persona, appropriatezza ed efficacia delle cure erogate e l'offerta dei servizi ostetrici e pediatrici-neonatologici nella rete regionale. Il secondo punto dell'accordo prevede l'umanizzazione dell'evento nascita per effetto del miglioramento dell'assistenza ostetrico e pediatrica-neonatologica, l'espletamento del parto indolore, l'allattamento materno precoce e il *rooming-in*. La Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha predisposto il documento "Controllo del dolore durante il travaglio ed il parto vaginale tramite procedure analgesiche", con il quale si sono volute definire le modalità operative per praticare l'analgesia nel quadro di un articolato programma di assistenza alla gravidanza, in accordo con i princìpi espressi nell'ambito del Piano sanitario nazionale 2006-2008. E' fondamentale, quindi, individuare e condividere, a livello nazionale e regionale, le regole con le quali le diverse professionalità operanti nel sistema si possono confrontare, sulla base delle rispettive competenze. Il dolore fisiologico del parto va inteso come condizione dolorosa diversa da quella conseguente a condizioni patologiche. La gravidanza - è stato ricordato anche in quest'Aula - non è una condizione patologica. come peraltro ogni preparazione al parto, dovrebbe far parte di un programma di assistenza alla gravidanza, inteso come globalità del nascere, e non piuttosto come evento isolato, spesso oggetto di scarsa informazione, proposta solo in sala parto. Vorrei ricordare che non sempre l'analgesia epidurale è l'intervento di controllo del dolore più appropriato. Fra l'altro, ha effetti sull'allattamento al seno.

da questo punto di vista, che ha un'alta percentuale di parti fisiologici e persino di parti a domicilio. Lo stesso accordo prevede la riduzione della mortalità neonatale e materna, ottimizzando il numero dei reparti pediatrici e dei punti nascita (con la riduzione del numero di punti nascita con meno di 500 parti parti l'anno), concentrando le gravidanze a rischio, programmando per tempo l'ingresso della partoriente in una struttura di terzo livello e prevedendo inoltre nei punti nascita una guardia medico-ostetrica e pediatrico-neonatologica, attiva 24 ore su 24. In tutto il percorso assistenziale un'attenzione particolare deve essere posta alla sempre maggiore presenza di donne straniere, soprattutto extracomunitarie, alle quali deve essere garantita la comunicazione interculturale e l'assistenza specialistica per i soggetti affetti da mutilazioni genitali. Il quarto punto dell'accordo già citato prevede che debba essere favorito il trasporto neonatale, quale componente essenziale di un piano di regionalizzazione delle cure perinatali. Il Ministero intende inoltre prevedere la sperimentazione di un progetto sull'implementazione di percorsi clinico-organizzativi integrati per la promozione dell'appropriatezza nel percorso nascita e la riduzione della pratica del taglio cesareo. Per quanto riguarda la salute dei bambini fin dai primi mesi di vita, si segnala che questa è stata più volte oggetto di iniziative di informazione e sensibilizzazione da parte di questo Ministero. Ci si riferisce in particolare alla campagna «Genitori più» (realizzata in collaborazione con la Regione Veneto, la Federazione italiana dei medici pediatri e l'UNICEF), avente la finalità di portare a conoscenza dei genitori alcune semplici azioni, da attuare autonomamente, di dimostrata efficacia per prevenire malattie, malformazioni, infezioni, traumi, incidenti, ma anche difficoltà cognitive e relazionali del nascituro. Inoltre, per promuovere l'allattamento al seno, il 6 aprile 2009 si è insediato presso il nostro Ministero il Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento al seno. Va però sottolineato che la maggior parte delle misure proposte nelle mozioni in esame appartengono alla diretta competenza regionale, come previsto dall'attuale quadro normativo di livello costituzionale, e pertanto l'azione del Governo può espletarsi solo con la forma dell'invito e del sollecito agli organi regionali competenti. Inoltre, le maggiori risorse da destinare all'implementazione dell'anestesia epidurale negli ospedali dovrebbero derivare da interventi di razionalizzazione ed efficientamento delle attività ospedaliere, i quali devono essere realizzati dalle autorità regionali, in particolare mediante la riconversione dei punti nascita sotto i 500 parti.

le parole: «ad intraprendere azioni al fine di promuovere l'assegnazione» con le seguenti: «ad intraprendere azioni al fine di garantire le procedure analgesiche nel corso del travaglio del parto vaginale nelle strutture individuate dalle Regioni all'interno di apposito programma». Questo in coerenza con la formulazione adoperata nei nuovi LEA e condivisa con le Regioni.

Grazie! Se non la garantisce la può pure promuovere! Tutto questo quando la sua maggioranza è assente dall'Aula e a garantire un minimo di presenza a questo dibattito c'è solo l'opposizione.

Il parto cesareo dovrebbe essere una soluzione quando non può espletarsi un parto fisiologico, ma non è più così. L'argomento che voglio sottolineare con il mio intervento è che il parto è un evento fisiologico

e all'aumento dei parti cesarei. Perché è aumentato oltre i limiti ragionevoli il ricorso al parto cesareo? Perché questa disparità tra le varie Regioni? Molto è stato detto e non voglio riprendere tutti gli argomenti, ma vorrei sottolineare

la necessità di una definizione più precisa di questi due ruoli. Il secondo aspetto che voglio sottolineare è il numero di contenziosi sul

bisogna riportare il parto nella dimensione di un evento fisiologico e lavorare per questo. Laddove, invece, questa realtà viene medicalizzata diventa facilmente

per questi percorsi-parto in cui l'ostetrica è la figura centrale. sul tema della maternità e del parto ci sono tante differenti posizioni e teorie, dalla difesa del parto come evento primordiale e naturale, e quindi tale da non richiedere alcuna interferenza esterna, a quello del parto ipermedicalizzato, il cesareo programmato, anche quando la salute della mamma e del bambino non lo richiedano, praticato e diffuso soprattutto nelle cliniche private, spesso con l'unico scopo di un maggiore guadagno. Su una cosa penso però che oggi, nel 2009, dobbiamo essere tutti d'accordo, e cioè nel riconoscere alle donne, in questo momento particolare della loro vita, una serie di diritti irrinunciabili, tra cui quello fondamentale di poter scegliere consapevolmente come far venire al mondo il proprio figlio. Ma perché questo sia possibile è necessario che alle donne siano dati tutti gli strumenti per poter scegliere: tutte le informazioni sul parto naturale e i vari tipi di parto naturale, sulle eventuali pratiche analgesiche disponibili e le loro conseguenze, sul parto cesareo e gli eventuali rischi conseguenti per la mamma e il bambino. L'eccessiva medicalizzazione della maternità ha portato la società a vedere nel parto una patologia da curare e nella donna in stato di gravidanza un malato da monitorare. si sono moltiplicate le analisi di diagnosi prenatale con strumenti sempre più sofisticati, che spesso superano di gran lunga il numero consigliato, e i parti cesari. Tutto ciò ha tolto alle donne il ruolo centrale che invece hanno in questo evento, anche perché non c'è nascita senza un'accoglienza da parte della donna e senza una simbiosi madre-bambino. Le statistiche indicano che le donne più consapevoli e più informate sono in grado di non farsi influenzare troppo dalla pratica medica e dall'ambiente e sanno far valere la propria volontà nel gestire le cure, limitando gli eccessi, in sintonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Allora direi che è importante ridare alla donna e al suo senso di responsabilità l'ultima parola. L'articolo 32 della Costituzione - come ho già sottolineato durante il dibattito - sancisce che è compito dello Stato garantire la salute della popolazione. Una sanità pubblica degna di un Paese che si dice civile deve fare in modo che a tutte le donne, indipendentemente dalle condizioni sociali, vengano dati uguali diritti: diritto alla salute della madre e del bambino, diritto ad un parto consapevole nel rispetto dei propri tempi e delle proprie necessità, diritto all'assistenza psicofisica *pre* e *post partum*, diritto ad avere tutte le informazioni sui rischi e le conseguenze del parto di cui la donna sarà protagonista. Visto che siamo nel terzo millennio, cerchiamo di evitare che la frase biblica «tu donna partorirai nel dolore» diventi una condanna, ma che sia eventualmente una scelta, e di fare in modo che l'epidurale, per coloro che vogliono farne uso, sia garantita e gratuita; facciamo in modo che non siano calcoli meramente economici a dettare i tempi e i modi della maternità e del parto. Se vogliamo realmente difendere la famiglia e se - come dice l'Organizzazione mondiale della sanità la venuta alla luce di un bambino in una famiglia, nucleare o estesa, è la fase di estensione del ciclo vitale della stessa, è dalla salvaguardia di questo primo nucleo

ed era previsto che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, il Ministro del lavoro avrebbe emanato un decreto per dare attuazione a questo fondo a tutela dei lavoratori. Purtroppo quel termine è scaduto da un anno e non abbiamo avuto risposta, nonostante un'interrogazione che abbiamo presentato con la collega Fontana ed altri senatori

Poiché arrivano richieste al Ministero del lavoro e della salute per avere notizie sul Fondo per le vittime dell'amianto e queste richieste vengono continuamente dirottate dalla segreteria del Ministro alla Direzione generale per le politiche previdenziali, alla Direzione generale tecnologia e comunicazione, alla Direzione generale tutela delle condizioni del lavoro, credo che sarebbe buona cosa per il Governo dare risposta alle esigenze dei lavoratori che hanno subito gravissime patologie da amianto e non prenderli in giro. Sono passati oltre sei mesi, è scaduto un termine da un anno ed i lavoratori colpiti dall'amianto stanno aspettando una risposta da questo Governo e dai Sottosegretari interessati alle questioni relative alla salute.

in discussione generale. Ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi dei colleghi e ricordo che, per quanto riguarda i dispositivi delle mozioni, non dobbiamo mai dimenticarci che la parte preponderante della responsabilità della politica sanitaria è ormai stata

è chiaro che quella del Governo può essere soltanto un'azione di controllo e d'indirizzo, ma non può essere impegnativa per le Regioni stesse. Detto questo, il voto del Gruppo della Lega Nord è favorevole a tutte le mozioni presentate.

gravido - per usare una terminologia adeguata - di buone cose. Le tre mozioni hanno portato in Aula un tema di grande interesse, interesse, con un linguaggio comune, com'è stato rilevato. Vorrei soltanto trattenere per me, allo scopo di sottolinearle in una dichiarazione di voto, naturalmente favorevole, per le tre mozioni,

essenziale: basterebbe andare a guardarne la definizione non su un testo di ostetricia o ginecologia, ma sul sito di Wikipedia, per sapere quali sono le indicazioni per un parto cesareo e quali no. Trattengo poi il termine

nelle strutture competenti, la competenza dei professionisti può essere più sicura e certa e problemi riferiti alla medicina difensiva e al contenzioso vengono meno. Basti ricordare che negli Stati Uniti, che sono la patria del contenzioso e della medicina difensiva, la percentuale dei parti cesarei è di gran lunga inferiore alla nostra. La terza parola che trattengo per me è «dati»: i dati non sono pochi né assenti, ma devono essere utilizzati in maniera intelligente. Esiste una medicina basata sull'evidenza, perciò dovrebbe esistere anche un'organizzazione basata sull'evidenza.

rilevo sempre che il dato più significativo è che il Governo ha chiesto di tradurre alcune azioni che venivano richieste in intenzioni. Vi sono sicuramente motivi che riguardano l'assetto federale della sanità del nostro Paese: in questo, credo si possa riscontrare anche un limite, ma il Governo non dovrebbe tuttavia sottrarsi alla responsabilità di assumere per sé quel che deve. L'inserimento nei LEA del parto indolore è un'azione che compete al Governo.

dell'andamento dei lavori, di tutte le considerazioni intelligenti, pacate e costruttive che sono state fatte in questa discussione nell'analisi delle tre mozioni. Il

la preoccupazione dell'offrire e del garantire è assolutamente inserita nell'alveo di una programmazione con le Regioni. È ovvio che ogni Regione deciderà dove allocare i punti di riferimento nei quali si garantirà

Mi dispiace ribadire a chi in questo momento si sta sbracciando per dire no, che il Titolo V della Costituzione alloca la responsabilità alle Regioni per poter programmare i servizi territoriali;

a titolo gratuito e garantita. Ciò non si può fare, chiaramente, in tutti gli ospedali italiani. Mi dispiace molto - lo devo dire al termine della mia dichiarazione di voto - che una collega che reputo intelligente e soprattutto molto preparata,

perché soltanto con il ragionamento, la pacatezza, la volontà propositiva, con un intendimento continuo e costante, soprattutto da parte delle donne (perché spesso e volentieri sono proprio le donne che creano i più grandi ostacoli a se

per rassicurare le senatrici che hanno espresso alcuni dubbi sulla riformulazione richiesta alla mozione

chiedo di mantenere «le prestazioni garantite a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza», aggiungendo la formulazione, che abbiamo

a qualche risultato. Non parteciperò al voto perché è stato detto che le mozioni non impegnano il Governo. Va bene che impegnano le nostre ore in attesa del *rais* che viene a parlare domani mattina, ma non si riesce a capire a cosa servono le mozioni se nel dispositivo non si impegna il Governo.

ritiro della sua firma. Prima di passare alla votazione delle mozioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Signor Presidente, nella fase conclusiva dei nostri lavori di ieri era stato avanzato l'auspicio da parte del senatore Divina che si riprendesse in considerazione la decisione

affinché si prenda in considerazione l'opportunità di dare questo palco - ricordo ancora una volta - concesso esclusivamente al re Juan Carlos e a Kofi Annan per far parlare qualcuno che non conosce né pratica la democrazia. Se si ritiene assolutamente fondamentale concedere quest'Aula, visto e considerato che anche nella Conferenza dei Capigruppo non vi è stata l'unanimità, grazie all'opposizione del Gruppo dell'Italia dei Valori - Emma Bonino assente perché impegnata in una conferenza contro la pena di porte nella Repubblica democratica del Congo - almeno, in apertura dei lavori della seduta pomeridiana, se ne possa discutere ed arrivare ad un voto. Concedere un'Aula quando non vi è unanimità,

anch'io intendo annunciare lo sciopero della fame come forma non di protesta, ma di proposta e di dialogo con la Presidenza del Senato. Tengo a sottolineare la situazione imbarazzante che si sta venendo a creare: l'istituzione Senato sconvoca una seduta dell'Assemblea per ospitare l'intervento del Presidente dell'Unione Africana

visto che si ospita un intervento esterno, saremo una sorta di sala congressi. La situazione imbarazzante è che il Senato invita il Presidente dell'Unione Africana

il premier Berlusconi ha inventato la solita scusa per non andare a Ciampino ad

Poretti, ad un incidente internazionale se Gheddafi verrà in quest'Aula. Un piccolo inciso: non abbiamo fatto parlare in quest'Aula

Signor Presidente, non parlerò di Gheddafi, ma del saccheggio che subisce il popolo degli Ogoni nel Delta del Niger. Domenica scorsa la ha documentato la violazione dei diritti umani e i gravissimi danni ambientali di cui sono responsabili le compagnie petrolifere, incluse ENI, AGIP e SNAM Rete Gas, nel Delta del Niger. La responsabilità di tali compagnie nelle violazioni dei diritti umani e nei dissesti ambientali è dimostrata proprio per loro diretta ammissione. Ieri un dispaccio dell'agenzia di stampa APCOM ci ha informato che la Shell la Shell ha accettato di pagare 15,5 milioni di dollari per evitare di comparire in un clamoroso processo per la morte di Ken Saro-Wiwa, ucciso il 10 dicembre 1995 insieme ad altri otto attivisti.

battevano contro i danni ambientali causati dalle attività petrolifere della Shell e delle altre multinazionali nel Delta del Niger e contro la miseria e l'arretratezza a cui il Governo nigeriano condannava il suo popolo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Gruppo dell'Italia dei Valori è doveroso ricordare nelle istituzioni quegli uomini che si battono contro la violenza delle multinazionali e dei grandi potentati per liberare i loro popoli dall'oppressione e affrancarli dalla miseria.